Grazie

"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Onorevoli colleghi, informo che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere sul disegno di legge in materia di riconoscimento della lingua italiana dei segni e che la Commissione giustizia non ha concluso l'esame dei disegni di legge sul codice antimafia. Informo inoltre che il relatore Tomaselli ha chiesto di poter anticipare l'esame dei disegni di legge sulle politiche spaziali e aerospaziali.

nn. 1110, 1410 e 1544. I relatori, senatori Pelino e Tomaselli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il disegno di legge al nostro esame ha lo scopo dichiarato, all'articolo 1, di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana, l'ASI, attribuendo al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali nell'interesse dello Stato. è il frutto di un lavoro istruttorio importante. Si partiva da tre disegni di legge che si ponevano la comune esigenza di riformare il ruolo dell'Agenzia spaziale italiana, collocando una maggiore attenzione allo sviluppo industriale del comparto spaziale nazionale. A tale scopo, in Commissione industria sono state sentite le principali associazioni del settore spaziale e aerospaziale, che hanno rappresentato le proprie esperienze in proposito, di cui questo testo ha certamente tenuto conto. Nel merito, brevemente, l'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di indirizzo governativo e il coordinamento delle politiche concernenti, appunto, il settore spaziale e aerospaziale. L'articolo 2 stabilisce che per tali compiti il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un apposito Comitato, composto da diversi Ministri che, a vario titolo, sono competenti in materia. Le competenze del Comitato sono elencate in forma analitica al comma 6 dello stesso articolo 2. L'articolo 3 stabilisce una serie di norme e di modifiche per favorire il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, mentre l'articolo 4 apporta le necessarie modifiche allo statuto dell'ASI, l'Agenzia spaziale italiana. Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono disposizioni transitorie e di coordinamento e le necessarie abrogazioni. L'ASI, istituita quasi trenta anni or sono, nel 1988, è già stata riordinata con il decreto legislativo n. 128 del 2003. Nel maggio 2011 ha visto un ulteriore riassetto per effetto del decreto legislativo n. 213 del 2009. Quel decreto, tra le altre cose, stabiliva l'autonomia statutaria degli enti di ricerca. L'Italia si è quindi dotata per tempo degli strumenti per governare un settore e per programmare sin dal 1988, attraverso dei piani triennali, strumenti idonei a garantire la gestione e la stabilità dei finanziamenti. Dobbiamo evidenziare che l'Italia è sempre stata all'avanguardia in questo settore, contraddistinto da programmi di grande complessità tecnologica e organizzativa, con costi elevati, e di durata pluriennale, coinvolgenti molteplici accordi di cooperazione internazionale. Oggi, queste caratteristiche si scontrano con un contesto economico internazionale sempre più difficile. Ma voglio ricordare che lo spazio rappresenta un settore importantissimo, con importanti ricadute nello sviluppo dell'economia e nella crescita del nostro Paese. In generale, ogni scoperta generata dalla ricerca nel settore aerospaziale crea innovazione negli altri settori industriali ad esso collegati, che si concretizza nella produzione di oggetti utili nella vita di tutti i giorni. Vorrei solo ricordare gli effetti che la ricerca aerospaziale produce nel mercato delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare, ma anche delle applicazioni nel campo delle osservazioni della Terra. Lo spazio va quindi considerato un sistema complesso per le conoscenze, i settori industriali, le applicazioni e gli utenti globalmente coinvolti. Allo stesso tempo esso si sviluppa, da sempre, tramite un cospicuo numero di cooperazioni e di *partnership* internazionali, sia nel settore della ricerca, che nel settore industriale che da esso discende. Va rilevato che la disciplina che ha regolato l'Agenzia spaziale italiana in questi anni ha sempre anticipato e agevolato le attività proprie nel campo spaziale. In questi anni essa è stata incaricata di realizzare i piani approvati dal Governo e ha interagito con le corrispondenti Agenzie degli altri Paesi, avendo un ruolo istituzionale e funzionale di ente di ricerca, limite che non aiuta a far cogliere pienamente all'Italia le opportunità internazionali e le potenzialità applicative del settore. Per il tramite dell'ASI, l'Italia ha oggi un ruolo di primissimo piano, in campo internazionale e a livello europeo, dov'è stabilmente il terzo Paese per contribuzione e presenza nei programmi dell'ESA, l'Agenzia spaziale europea. A livello mondiale è, invece, ormai consolidata la collaborazione con la NASA, la National aeronautics and space administration, nell'ambito di importanti missioni scientifiche e interplanetarie e soprattutto per la partecipazione allo sviluppo della stazione spaziale internazionale (un'alta percentuale dei moduli abitati e dei componenti sono stati realizzati dalla nostra industria nazionale) e alle missioni degli astronauti italiani. Va ricordato che le aree tecnologiche che rappresentano i punti di forza dello spazio in Italia sono molteplici: lo sviluppo di satelliti per telecomunicazioni, di satelliti scientifici, di satelliti di osservazione *radar*, di moduli pressurizzati abitati e di sistemi di propulsione e di lancio. Mediamente, negli anni una percentuale prossima al 75 per cento degli investimenti gestiti dall'ASI ha riguardato progetti a valenza industriale e applicativa e questo per effetto delle approvazioni dei piani triennali spaziali, cioè di un opportuno governo del settore. Grazie al continuo progresso delle sue attività, sempre più indirizzate alle applicazioni dello spazio, la stessa Agenzia spaziale italiana ha assunto negli anni una configurazione istituzionale che l'ha portata ad operare concrete e fattive integrazioni con altri settori della pubblica amministrazione, con enti pubblici centrali e territoriali. Questa evoluzione del ruolo dell'ASI si è concretizzata anche grazie all'utilizzo di risorse finanziarie - quali ad esempio i trasferimenti dell'amministrazione della Difesa - complementari a quelle previste nel bilancio ordinario dell'ente, che - va ricordato - è a carico del Fondo ordinario per il finanziamento nazionale degli enti di ricerca. Il ruolo dell'Agenzia si esplica anche attraverso diverse società controllate o di cui fa parte, come Altea (servizi ingegneristici e logistici), CIRA (Consorzio italiano di ricerche aerospaziali), e-Geos (società per la promozione e lo sviluppo del mercato nazionale ed internazionale delle applicazioni e dei servizi commerciali nel settore dell'osservazione della Terra), Elv spa (società nel settore dell'industria aerospaziale). Il presente disegno di legge , proprio per il complesso della materia trattata e degli interessi coinvolti,

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di alta direzione politica e di vigilanza del settore. Allo stesso modo viene assegnata un'apposita delega ad un Sottosegretario per le politiche spaziali e aerospaziali. Si tratta insomma di un complesso di nuove norme, che giudichiamo veramente positive per la *governance* del settore spaziale e dell'aerospazio e di cui chiediamo l'approvazione all'Assemblea del Senato.

Il provvedimento è volto infatti a conferire maggiore centralità alle politiche spaziali e aerospaziali del nostro Paese, il quale vanta da sempre una posizione di *leadership* a livello mondiale nel settore, rappresentando

L'importanza di questa filiera non deriva però soltanto dal contributo che essa può garantire in termini di occupazione e di valore aggiunto, ma anche dal fatto che essa integra e promuove lo sviluppo di competenze, di processi e di tecnologie vitali per l'economia nel suo complesso e sempre di più per la vita quotidiana di ciascuno di noi. Gli sforzi nel settore spaziale e aerospaziale, al fine di garantire il raggiungimento dei rigidi *standard* richiesti,

sia nei centri di ricerca pubblici e privati che nelle stesse università del nostro Paese. Il comparto rappresenta uno dei tasselli fondamentali nel quadro delle alte tecnologie dove industria, università e comunità scientifica italiane sono riuscite a consolidare una posizione di rilievo nel quadro internazionale, sviluppando straordinarie e importanti eccellenze. In una prospettiva di crescita del Paese non si può, quindi, prescindere dalla salvaguardia e valorizzazione di questo settore che oggi rappresenta un tassello fondamentale per l'innovazione nell'industria e nel sistema economico nazionale, oltre che in tema più tradizionale di sicurezza e difesa. La necessità di riorganizzare questo comparto nasce, da un lato, dai profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi trenta anni, mai del tutto recepiti a livello normativo e legislativo,

e, dall'altro lato, dal fatto che le attività spaziali e aerospaziali coinvolgono molteplici settori sotto la competenza di diversi Ministeri.

che guardi a industria, difesa, ambiente, ricerca, trasporti, agricoltura, vocazioni regionali e politiche comunitarie, al fine di garantire un coordinamento il più possibile completo ed efficace delle politiche del settore.

che darà una cornice normativa a una prassi positiva che ha determinato risultati importanti - ce lo hanno confermato sia gli attori istituzionali che i rappresentanti del vasto mondo delle grande e piccole imprese, che hanno potuto godere di questa *governance* unitaria - sia nel coordinamento delle politiche a livello nazionale, sia nel convogliare imprese, sistemi industriali e i vari Ministeri coinvolti in un unico lavoro comune.

sforzo significativo e sempre più vincente dal punto di vista degli interessi nazionali che la stessa Agenzia spaziale italiana va compiendo negli ultimi anni sia in Italia che a livello comunitario e globale. Indubbiamente, la riforma di questo settore porterà ricadute positive sull'industria e sulle piccole e medie imprese operanti nel settore. Nella nuova prospettiva, tra i principali obiettivi del comitato interministeriale vi è la definizione e l'incentivazione di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche sia nazionali, comunitarie che regionali (spesso non coordinate tra loro) e il mondo dell'impresa; la determinazione delle priorità di ricerca e degli investimenti pubblici del settore al fine di diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché quello di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese. lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica, nonché dovrà favorire il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni. La continuità stessa dell'Agenzia spaziale italiana è, infatti, il presupposto e il cardine inderogabile su cui si basa questo lavoro per garantire la prosecuzione dei programmi spaziali in atto e per una strategia ancora più chiara e vincente per lo sviluppo dell'industria spaziale in Italia. Non a caso l'ASI, anche tramite la propria partecipazione al comitato interministeriale, assurgerà a soggetto fondamentale in termini di *governance* generale del sistema, fungendo da raccordo tra il sistema industriale e della ricerca e tutte le istituzioni nazionali e internazionali. Infine, signora Presidente, colleghi, ricordo come la stessa Commissione europea, con la sua comunicazione dell'aprile 2011, definiva la strategia spaziale della stessa Unione a servizio dei cittadini europei come fondamentale. A tal riguardo venivano indicati tre obiettivi: il primo di carattere sociale, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa - dice la Commissione europea - in ambiti quali l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell'informazione. ricadute nel campo economico, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d'innovazione, contribuendo alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione. sono le ricadute di ordine strategico, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell'Unione sulla scena mondiale e a contribuire alla sua indipendenza economica e politica. Vi sono, in queste parole della comunicazione della Commissione europea dell'aprile 2011, forse gli aspetti più significativi di questo ambizioso lavoro che anche nel nostro Paese si sta portando avanti negli ultimi anni e che oggi trova un suo suggello istituzionale

ad una delle eccellenze più straordinarie del nostro Paese costruendo una *governance* non solo di primaria rilevanza da punto di vista politico-istituzionale affidandone la responsabilità alla principale autorità politico istituzionale del Paese, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, utile a dar autorevolezza a chi opera in tale settore e, nel contempo, si valorizza la caratteristica di fattore fondamentale per la crescita e la competitività dell'intero sistema Italia, di un comparto, quello dello spazio e dell'aerospazio, che con legittima ambizione vede oggi il nostro Paese in una posizione di *leadership* mondiale sia nella ricerca che nell'industria che nei servizi applicativi. Con queste norme le istituzioni, a cominciare da Governo e Parlamento, colleghi, suggellano tale importanza strategica e mettono le basi per ulteriori ed importanti successi del settore dell'aerospazio italiano nel mondo.

Signora Presidente, stiamo discutendo e affrontando un argomento strategico per il nostro Paese. La questione delle politiche spaziali e aerospaziali ha una grandissima rilevanza come hanno già ben delineato, nelle loro relazioni i colleghi Pelino e Tomaselli. Questo disegno di legge vuole assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana; per questo motivo, esso attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la direzione, la responsabilità di indirizzo politico e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali. Tutto ciò lo fa nell'interesse dello Stato, perché si tratta, com'è stato ben evidenziato, di un settore strategico. Verrà istituito quindi un Comitato interministeriale, una vera e propria cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che avrà precisi compiti di indirizzo e di coordinamento in materia spaziale e aerospaziale. La partecipazione dei diversi Ministeri interessati, molteplici (quasi tutti direi), dà il senso dell'interesse e della trasversalità di queste politiche: difesa, interno, beni e attività culturali e turismo, politiche agricole alimentari e forestali, istruzione università e ricerca, sviluppo economico, infrastrutture e trasporti, ambiente e tutela del territorio e del mare, affari esteri e cooperazione internazionale, economia e finanze. Quindi, una molteplicità di tematiche, tutte strettamente interrelate agli indirizzi e alle azioni concrete che il Comitato potrà direttamente orientare nei confronti di questi temi e interessi nazionali. Alla base c'è quindi la consapevolezza del rilievo e della strategicità delle politiche aerospaziali, che richiedono un coordinamento non sporadico e un approccio di sistema. Il Comitato, la cabina di regia, dovrà in primo luogo definire gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con riferimento alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle sue ricadute sul terreno produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del documento strategico di politica spaziale nazionale. Con il documento strategico si definiranno poi la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e e di servizi applicativi a favore della crescita economica del Paese. Fra i numerosi compiti del Comitato, ne voglio richiamare alcuni che mi appaiano particolarmente di rilievo: definire le priorità di ricerca e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi; definire il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali, perseguendo le indispensabili sinergie fra risorse pubbliche e private destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali. La questione delle sinergie fra risorse pubbliche e private, che qui vediamo in relazione al settore spaziale e aerospaziale, riterrei debba essere un filo conduttore anche per quanto riguarda altri settori strategici strategici del nostro Paese e, in generale, nel campo della ricerca. Un altro compito che sarà affidato alla cabina di regia è quello di promuovere, sulla base delle esigenze condivise dalle amministrazioni interessate, accordi di programma che prevedano il finanziamento, da parte dei diversi Ministeri interessati, di servizi applicativi, sistemi e infrastrutture spaziali. Vorrei sottolineare il fatto che, nell'elaborare le linee strategiche, la cabina di regia dovrà favorire lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese e promuovere il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto Il Comitato interministeriale svolgerà poi compiti importanti in relazione all'Agenzia spaziale italiana, come ha ben ricordato la senatrice Pelino: in questo campo avrà compiti di indirizzo e supporto per la definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali, assicurando il coordinamento dei programmi dell'Agenzia con le attività delle amministrazioni sia centrali che periferiche. L'Agenzia è stata istituita con grande intuizione quasi trent'anni fa, nel 1988, e nel 2009 è stata inclusa da un decreto legislativo tra gli enti di ricerca consentendogli così di operare nel contesto scientifico e industriale, stando al passo con le agenzie aerospaziali di altri Paesi. C'è poi, nel provvedimento in esame, un altro tema è prevista la valutazione complessiva dei risultati ottenuti dai programmi, dei ritorni in termini strategici ed economici, ma anche delle sue ricadute per gli aspetti sociali. Entro il 30 giugno di ogni anno il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale dovrà predisporre una relazione alle Camere con l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale. Il Parlamento avrà così la possibilità e la responsabilità di valutare e richiedere al Governo, se necessario, di riorientare le politiche e gli indirizzi dati.

dei lanci di satelliti, come Ariane e Vega, o della partecipazione italiana all'utilizzo della Stazione spaziale internazionale da parte dei nostri straordinari astronauti, come Samantha Cristoforetti. Queste vicende, note al grande pubblico, non sono che la punta di diamante di una vasta, articolata esperienza e competenza italiana in questo campo, sia nel versante della ricerca che in quello industriale. Per essere competitivi sono due le questioni che abbiamo davanti, entrambe cruciali e assolutamente complementari: la prima è quella della ricerca; la seconda è quella del trasferimento dei suoi risultati. Dobbiamo essere capaci di raccogliere gli straordinari risultati della ricerca italiana e ben indirizzare la sua spinta alla innovazione tecnologica per valorizzarla a livello industriale. Strategico è il tema della ricerca. L'ha capito bene la mia Regione, l'Emilia-Romagna, che l'ha affrontato con la realizzazione dei tecnopoli e della rete ad alta tecnologia. Nella mia realtà provinciale è stato realizzato, ad esempio, un tecnopolo con competenza specifica in campo aerospaziale che può fornire una ricerca molto avanzata in tema di tecnologie aeronautiche e satellitari. Anche nei territori esistono quindi grandi competenze nella ricerca, così come sono presenti imprese piccole e medie anni hanno saputo innovarsi, riuscendo a competere in un mercato sempre più globalizzato e competitivo. È quindi molto importante che la cabina di regia sulle politiche aerospaziali conosca anche queste realtà, che possono contribuire in modo significativo alla crescita e allo sviluppo della ricerca e dell'industria italiana. dell'industria italiana. Sono in particolare le piccole e medie imprese che vanno supportate ed aiutate per superare gli ostacoli che derivano dalle loro dimensioni che ne limitano la possibilità di investire direttamente in ricerca e innovazione e di competere sui mercati internazionali. Per questo è molto importante che la ricerca venga indirizzata alle loro esigenze, quelle delle piccole e medie imprese italiane. L'industria italiana è la quarta in Europa e la settima nel mondo in questo settore. Anche negli anni della crisi economica l'industria aerospaziale italiana ha continuato a crescere. Basti ricordare che dal 2008 il fatturato del settore ha avuto un incremento del 43 per cento, con ricavi per 13 miliardi di euro, di cui 7 miliardi derivanti dall'*export*. un settore strategico, quindi, in termini economici e occupazionali, come hanno bene evidenziato i relatori nella loro illustrazione del provvedimento. Un settore strategico anche per le straordinarie ricadute che questo settore ha su altri settori: che Internet, questa straordinaria invenzione e innovazione del nostro mondo, deriva proprio dalla ricerca in campo aerospaziale. Le implicazioni, quindi, della ricerca in questo campo e le sue ricadute sono molteplici. Non a caso stiamo assistendo, ad esempio, al rapido sviluppo nel settore dei satelliti ad alto livello di integrazione.

non solo grandi possibilità e potenzialità, ma le condizioni concrete per competere in un settore strategico che cambierà nel corso dei prossimi anni il panorama del settore spaziale nazionale ed internazionale, con tecnologie che che potranno permettere la radicale riduzione dei costi ed il miglioramento della qualità dei servizio in molteplici aspetti della nostra vita quotidiana. Si tratta, fra l'altro, di innovazioni tecnologiche che potranno essere particolarmente adatte alla partecipazione delle piccole e medie imprese ad alto contenuto tecnologico. Con questa cabina di regia, la nostra filiera nazionale spaziale ed aerospaziale, già molto rilevante, avrà ancora di più la possibilità di svilupparsi in modo competitivo e di partecipare ad una crescita economica del nostro Paese molto importante in termini economici, occupazionali

speriamo possa essere approvato da entrambe le Camere in tempi rapidi.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, sin dai primi anni Sessanta la politica spaziale ha avuto una notevole valenza strategica per il nostro Paese ed è grazie ad un bacino di eccellenza industriale, scientifica e tecnologica che l'Italia è una delle principali potenze spaziali d'Europa. Questo è avvenuto perché in primo luogo le attività spaziali italiane sono venute a svilupparsi nell'ambito di accordi e collaborazioni tra enti ed istituzioni come il Consiglio nazionale delle delle ricerche, l'Università di Roma e l'Aeronautica militare e, in secondo luogo, perché i modelli di cooperazione internazionale, che si sono rivelati particolarmente efficaci, hanno dato ottimi frutti, in in particolare i *partner* dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) hanno collaborato molto con l'Agenzia spaziale europea (ESA) e con la NASA stessa. Lo stesso Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, presentato nell'aprile 2015, ha identificato nello sviluppo del settore spaziale un'importanza strategica che richiede specifiche capacità anche nello studio, nella ricerca e nella realizzazione dei componenti. In questo quadro globale, lo spazio ha una sua caratterizzazione negli *standard* dell'industria internazionale. I dati economici sono molto frammentati e rendono difficile un'analisi sistematica dell'impatto socio-economico del settore. Sta di fatto, però, che il valore a livello globale, dai calcoli fatti, oscilla tra i 250 ed i 300 miliardi di dollari, cifre che sembrerebbero anche relativamente basse, se confrontate con i 300 miliardi delle *utility* italiane. Il PIL che fa riferimento al servizio spaziale ed aerospaziale è anche e soprattutto una fonte di fatturato indiretto per le tante aziende che sono in grado di produrre in questo campo. In tutto questo si inserisce il disegno di legge n. 1110 - ringrazio la senatrice Pelino qui presente - che ha la finalità di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali ed aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana. Tutto questo avverrà con l'attribuzione al Capo del Governo dell'alta direzione, della responsabilità politica generale e del coordinamento delle politiche dei Ministri relative ai programmi spaziali e aerospaziali nell'interesse dello Stato. Istituisce altresì un Comitato interministeriale con il compito di definire gli indirizzi del Governo, con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo,

appunto, insieme all'industria italiana, sempre attraverso gli investimenti istituzionali, hanno continuamente sviluppato una tradizione di alta tecnologia spaziale, anche propulsiva. politica spaziale per le nostre aziende e per il PIL nazionale, che la stessa Europa l'ha posta al centro della strategia europea 2020 e della nuova rivoluzione industriale.

nazionale. L'autonomia dell'ASI nel definire gli accordi bilaterali è pertanto una risorsa che consente all'Italia di avere opportunità scientifiche e industriali tali da posizionarsi meglio nei confronti dei *partner* europei.

rendendo coerenti e organici interventi settoriali, pur rilevanti, che in questi anni Governo e Parlamento avevano messo a punto. Il provvedimento mira a sviluppare il settore spazio e aerospazio, puntando uno specifico *focus* sulle piccole e medie imprese e sulla ricerca applicata e inoltre rende più netta e trasparente la gestione dell'Agenzia spaziale italiana.

anni hanno investito e difeso le aziende del settore e che presentano oggi tutte le carte in regola per contribuire al rilancio e allo sviluppo complessivo del settore, questa è sicuramente un'occasione da non perdere. Il disegno di legge in materia di politiche spaziali e aerospaziali

con i diversi organismi internazionali, definendo anche il quadro delle risorse finanziarie disponibili per il settore, perseguendo l'obiettivo di promuovere i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali e lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese. Anche il ruolo dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) viene amplificato e ne vengono valorizzate adeguatamente le competenze. L'ASI, anche tramite la partecipazione al Comitato interministeriale, assurgerà a soggetto fondamentale in termini di *governance* generale del sistema, fungendo da raccordo tra il sistema industriale e della ricerca e tutte le istituzioni nazionali e internazionali. Ritengo, infatti, che il futuro di tutto il comparto spaziale sia legato anche alla collaborazione internazionale e soprattutto ad una dimensione europea del settore. Il tema dello spazio e delle politiche spaziali rappresenta davvero oggi una grande opportunità per il sistema Paese. Si tratta di un settore che si basa su dinamiche interdisciplinari: a partire dalla ricerca, fino alle politiche industriali e tutto il mondo delle applicazioni. È per questo motivo che il disegno di legge mira ad assegnare alle politiche spaziali una *governance* quanto più unitaria e integrata. Un fatto importante poi è la definizione del quadro delle risorse finanziarie disponibili per il settore che necessita di investimenti significativi. l'ASI anche tramite la partecipazione al comitato interministeriale, assurgerà a soggetto fondamentale in termini di *governance* generale È noto a tutti infatti, che il futuro di tutto il comparto spaziale sia legato anche alla collaborazione internazionale e soprattutto ad una marcata dimensione europea del settore. Il disegno di legge punta al coordinamento delle politiche spaziali spaziali e aerospaziali con l'istituzione a Palazzo Chigi di un Comitato interministeriale *ad hoc*, presieduto dal Presidente del Consiglio; anche in questo c'è un chiaro salto di qualità. La finalità del disegno di legge è dichiarata nel primo articolo, quando si sostiene la necessità di «assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana». Il Presidente del Consiglio individuerà il Sottosegretario alla Presidenza con delega alle politiche spaziali e che potrà sostituirlo nel presiedere il Comitato composto da numerosi ed importanti Ministri. In relazione a specifici argomenti, potranno essere invitati alle sedute del Comitato anche rappresentanti di altri Dicasteri e di enti pubblici Comitato approva inoltre il documento strategico di politica spaziale nazionale, coordina l'attività dell'ASI con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche, individua le linee prioritarie, definisce gli indirizzi ancora, definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali e aerospaziali. Per svolgere i suoi compiti il Comitato si avvale del supporto tecnico dell'ASI e di eventuali esperti, gruppi di lavoro e comitati di studio. Lo sviluppo economico dell'Italia passa quindi, come affermato compiutamente dal relatore Tomaselli, anche per lo spazio. Ad ottobre 2016 è stata pubblicata la «Strategia spaziale per l'Europa». Alcuni tra i più importanti amministratori delegati del settore, penso a Donato Amoroso di Thales Alenia Space Italia, a Luigi Pasquali di Telespazio e a Giulio Ranzo di Avio, ne hanno discusso durante un evento, a cui ho avuto modo di partecipare, che ha visto anche la partecipazione dei ministri Calenda e

attraverso Altec, ha siglato un pacchetto di accordi industriali con Richard Branson per la costruzione in Italia di uno spazioporto da cui far partire navicelle per il turismo spaziale e per missioni scientifiche». Si aprono scenari di straordinaria importanza e il settore privato si sta muovendo con una rapidità esponenziale, soprattutto Oltreoceano. Dobbiamo innovare, quindi, usare le competenze e la capacità di pensiero e di lungimiranza di tanti nostri giovani ricercatori che nelle nostre università approfondiscono e studiano temi di così grande rilevanza. Lo fanno già negli Stati Uniti, in Cina e in India, e noi non siamo da meno, perché il nostro Paese, come veniva ricordato, è ai primi posti della classifica. Lo spazio sta muovendo verso nuove dimensioni. A partire dagli anni Cinquanta, quando i russi lanciarono il primo

è fatta di *big data*, e quelli satellitari rappresentano un bacino immenso di opportunità, spesse volte non considerate o sfruttate in modo solo parziale. Bisogna pertanto investire anche in nuove professionalità in grado di maneggiare ed elaborare dati, dare alla ricerca le giuste risorse per fornire all'industria una base evolutiva, che può essere cruciale per non perdere il passo con l'evoluzione. Non bisogna quindi sottovalutare tutta questa parte di ricerca e anche di *business*. In tale ambito - oggi è la giornata in cui Trump è in Italia non possiamo dimenticare i progetti NASA in questa stravagante epoca di Trump. Insomma, ci sono tante occasioni da non perdere, e il disegno di legge in discussione ci colloca nella dimensione di non perdere quantomeno nella riorganizzazione della *governance* e dei luoghi della decisione. Non è un caso che quando la terra nel 2009 tremò in Abruzzo e distrusse tanta parte della mia Provincia, colpendo aziende importanti come l'Alenia Spazio, ci rimboccammo tutti le maniche. Non potevamo perderla. A soli quattro anni dal terremoto che aveva distrutto il vecchio stabilimento e a soli due anni dalla posa della pietra del nuovo stabilimento, Thales Alenia Space ha inaugurato a L'Aquila uno dei più sicuri e moderni stabilimenti d'Europa.

competenti ingegneri di guardare al futuro. Stiamo inoltre organizzando il settimo distretto aerospaziale in Italia. Il disegno di legge in esame rappresenta quindi un ambizioso disegno di sviluppo, di rilancio economico e di creazione di nuovo lavoro; in tal modo i territori potranno organizzare e rafforzare le proprie potenzialità e potremo rendere l'intero settore più competitivo e proteso alla creazione di nuovo ed avanzato sviluppo.

collasserebbe il sistema delle telecomunicazioni; verrebbe meno la nostra capacità predittiva di eventi catastrofici, come ad esempio tempeste, tornado, cambiamenti climatici.

in altri settori come, ad esempio, i settori della salute, della medicina, del trasporto e della *computer* *science*. Questo si somma ai benefici che gli investimenti in ricerca e sviluppo già portano nel settore della conoscenza. Quindi oggi, signora Presidente, non è più sufficiente soltanto dire che lo spazio è un settore strategico ma dobbiamo dire che gli investimenti in questo settore creano posti di lavoro e contribuiscono a creare quell'economia europea competitiva e di altissimo livello che non si ritrova in altri settori. Non solo: le politiche spaziali danno agli Stati sovrani gli strumenti strategici necessari a creare le politiche nazionali. Quindi, signora Presidente, non è un caso che, ad oggi, vi siano sempre più Paesi che lanciano satelliti in orbita. Ad esempio, secondo i dati relativi al 2014, ci sono più di 50 Paesi che hanno un loro satellite in orbita

chiaramente ci dimostra che avere una politica spaziale riveste un ruolo strategico a livello globale. È importante mantenere un piede ben saldo nel campo aerospaziale perché ciò ci mette in condizioni di guidare tecnologie che, a loro volta, ci consentono di prendere decisioni strategiche per gli interessi nazionali del nostro Paese.

Grazie

In questo momento, a livello europeo, tale industria impiega 35.700 persone ed ha un *budget* totale di 6,5 miliardi di euro. La maggior parte di queste spese vengono fatte per programmi istituzionali più che programmi privati, quindi sono gli Stati

Luigi Broglio abbiamo aperto nel 1967 una base di lancio in Kenya, a Malindi, che abbiamo tutt'ora, anche se non è più usata per lanciare satelliti ma solo per fare telemetria degli stessi.

una partecipazione a maggioranza italiana e che contribuirà ad avanzamenti scientifici per quanto riguarda il pianeta rosso, Marte. Signora Presidente, ho esordito dicendo che oggi è un giorno storico perché il Parlamento parla di aerospazio. di aerospazio. Con questo disegno di legge abbiamo la possibilità di fare in modo che questa non sia l'ultima volta che il Parlamento parla di politiche spaziali, che abbiamo visto essere così importanti. Tuttavia, da questo punto di vista non posso che lamentarmi con i relatori per il fatto che, proprio tra i tre

signora Presidente, tutti gli altri Paesi europei si sono già attrezzati con organismi parlamentari stabili, che contribuiscono alla decisione proprio nel campo del monitoraggio e del controllo dell'attività governativa. Chiaramente,

che le hanno), che contribuiscono al dibattito sulla politica spaziale. Tanto è vero che esiste una Conferenza europea parlamentare sullo spazio,

spazio, e ho rilevato un passo indietro dell'Italia dal punto di vista parlamentare rispetto agli altri Paesi: non abbiamo un organismo parlamentare che possa presentarsi in quella Conferenza e sedersi ai tavoli per discutere della risoluzione che, nell'ambito di quell'assemblea,

fallito nel coinvolgere il Parlamento nelle decisioni di politica spaziale. Signora Presidente, reputiamo il disegno di legge in esame un provvedimento significativo. Esso prevede, infatti, l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio della direzione del coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali e, in particolare, istituisce un Comitato interministeriale con il compito di definire gli indirizzi del Governo

Il Comitato avrà il compito di indirizzare e supportare l'Agenzia spaziale italiana nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con i diversi organismi internazionali, definendo anche il quadro delle risorse finanziarie disponibili per il settore, perseguendo l'obiettivo di promuovere i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali e lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese. Siamo ben consci che il ruolo dell'ASI viene ampliato e ne vengono valorizzate le competenze, anche tramite la partecipazione al Comitato interministeriale, diventando soggetto fondamentale in termini di *governance* generale del sistema, con funzioni di raccordo tra il sistema industriale e della ricerca e tutte le istituzioni nazionali e internazionali. Tutto quello che va sotto il nome di aerospazio ha assunto un ruolo fondamentale a livello europeo e mondiale come motore di sviluppo e filiera di attività ad alto contenuto tecnologico, capace di produrre innovazione e generare effetti di catalizzazione e fertilizzazione su numerose aree industriali. Tutti i grandi Paesi industriali considerano il settore aerospaziale come un'area strategica in termini di valore economico. L'industria dell'aerospazio italiana si posiziona oggi nel complesso come quarto *player* in Europa e settimo nel mondo, con un fatturato di quasi 14 miliardi di euro nel 2014, secondo gli ultimi dati forniti dalla Operano nel comparto oltre 50.000 addetti, con investimenti in ricerca e sviluppo pari al 12 per cento dei fatturati, in linea con la media europea. Per quanto riguarda, in particolare, i prodotti e le tecnologie per lo spazio, l'industria italiana copre il 14 per cento delle attività europee, collocandosi al terzo posto

tra cui i grandi gruppi Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, Avio, Selex Galileo, oltre a tanti di piccole e "micro" dimensioni. sono 5.000, considerando solo le grandi aziende; tra gli 8.000 e i 9.000 includendo anche le attività operazionali e di logistica connesse. Voglio rivendicare anche il ruolo attivo che abbiamo avuto come Movimento 5 Stelle: finalmente l'Agenzia spaziale italiana sarà più trasparente e libera da politici riciclati e condannati. Siamo riusciti a far approvare in Commissione due importanti emendamenti anti-partitocratici. L'emendamento 3.5 prevede che il presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico dell'ASI «non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato» per i reati contro la pubblica amministrazione. Il secondo emendamento approvato, ovvero 33, l'A.S.I. è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale: *a)* le informazioni sull'attività complessivamente svolta; *b)* le informazioni sui *curricula* e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti; *c)* i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia». Sicuramente avremmo voluto qualcosa in più, in materia di scelta e funzioni del presidente dell'ASI: ai sensi della disposizione citata, il presidente si sarebbe potuto scegliere tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati operanti nel settore della ricerca, introducendo il requisito della riconosciuta onorabilità, così come previsto, a solo titolo di esempio, anche per i membri del consiglio di Certo vorremmo che si tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, come ci ha indicato il parere reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul provvedimento

tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, allo scopo di garantire il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo conseguentemente una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale. Vorremmo anche qui che, nei compiti, fosse più marcato, il fatto di promuovere il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni. Vorremmo far sì che venga che venga promosso il trasferimento di conoscenze, soprattutto nel settore della previsione e della prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo. Non ci convincono appieno alcune ambiguità, come quelle presenti nell'articolo 2, intitolato «Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale», quando si parla dello «sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica». troppo indistinto e ambiguo questo discorso tra civile e militare. Tutti noi sappiamo che l'industria aerospaziale possiede le caratteristiche per essere ascritta tra le attività produttive che si collocano a pieno titolo su un mercato completamente globalizzato. Nessun Paese avanzato può fare a meno di concorrere ad alimentarne la domanda di mercato, che non conosce alcun tipo di limitazione alla diffusione di natura geografica o culturale. Questi fattori, unitamente alla proprietà del settore di assorbire innovazione tecnologica da una pluralità particolarmente ampia di aree ingegneristiche, e quindi di fornitori di tecnologie, potrebbe far concludere che la localizzazione geografica dei sistemi produttivi in un'industria con un profilo spiccatamente internazionale sia poco rilevante. Al contrario, osserviamo una forte concentrazione del settore in un numero relativamente ristretto di aree geografiche, ma assistiamo anche alla nascita di organizzazioni e di sistemi per lo sviluppo delle attività industriali aerospaziali che comprendono la partecipazione congiunta di università, imprese e istituzioni impegnate in sinergia per far leva sulle capacità locali al fine di emergere nel mercato globale. Le applicazioni spaziali sono utili ad affrontare alcune delle più importanti sfide sociali e possono essere utilizzate nei settori più diversi, dalla tutela e monitoraggio dell'ambiente, all'agricoltura, dalla protezione civile alla salute dell'uomo e in numerosi altri contesti.

la relatrice Pelino e il relatore Tomaselli hanno fatto un lavoro veramente pregevole e credo che avrebbero meritato maggiore attenzione. Ho seguito attentamente le loro illustrazioni

negli anni ormai remoti si è sviluppata una capacità credibile di investimento, di produzione e di innovazione tecnologica straordinaria.

Nel nostro territorio si è sviluppata un'attenzione nei confronti delle eccellenze uscite dalle università, che probabilmente sarebbero state costrette ad andare all'estero o a trovare occupazioni di basso livello e, invece, hanno trovato un'occupazione di pregevole significato culturale e professionale. Ciò è molto importante.

dove c'è un interesse nazionale e, di fatto, uno sviluppo che va ben oltre il sistema spaziale e verso la ricerca. Quando si parla di ricerca duale, non c'è dubbio che si parla di ricerca a tutto campo e non solo nella direzione, ad esempio, del comparto difesa o altro. Di conseguenza, credo che gli investimenti fatti necessitino di maggiori risorse. Si sta facendo bene, ma si deve fare ancora meglio perché questi investimenti determinano occupazione in un settore di eccellenza che colloca il nostro Paese, come è stato ricordato, in un ruolo di primissimo livello nel contesto europeo e internazionale. Senza dubbio vanno premiate queste eccellenze che i territori hanno saputo sviluppare, vanno seguite e incentivate e in questo caso, seppure con una tardiva attenzione, il Senato, e in più generale il Parlamento, dovrà riservare loro attenzione. Muoviamoci, dunque, convintamente in questa direzione. Mi auguro che ci sia una condivisione ampia su questo tema, a dimostrazione che queste realtà non sono isolate ma sono attenzionate, sostenute e - lasciatemi dire - anche protette della politica nazionale, che deve di fatto assumersi questa responsabilità. *(Applausi

ancora una volta il Sud ad avere interesse affinché questo disegno di legge prenda piede e venga approvato. Il Mezzogiorno già da decenni patisce la mancanza di politiche industriali conseguente perdita di competitività da parte del sistema Italia ma, in particolare, con i drammi che la perdita di competitività impone a larghe fasce della nostra popolazione, particolarmente a quella meridionale, con perdita tragica, tragica, drammatica, di posti di lavoro. A questa perdita di posti di lavoro, ovviamente, va aggiunto un degrado terribile per quanto riguarda la

e arretratezze ataviche e, quindi, anche di potenziali capacità di intravedere futuro. con questo disegno di legge il Sud e, in particolare, l'impresa aerospaziale del Sud tornano a nutrire una speranza. Lo dico perché i poli aerospaziali di Campania e Puglia, particolarmente importanti e consolidati, troverebbero davvero una speranza nella risistemazione e nella rivisitazione delle funzioni che questo disegno di legge vuole dare ai vari attori che sono compresi nell'articolato di legge, a cominciare dalla istituzione del Comitato interministeriale. L'industria aerospaziale meridionale

il sistema della ricerca pubblica e privata, quella che è all'interno delle università, dei centri di ricerca, pubblici e privati, nonché tutto il sistema aeronautico che ha valenze sia militari che civili. scientifica italiana. Queste potrebbero essere considerazioni di buon auspicio affinché il disegno di legge trovi una larga adesione all'interno di questo Parlamento. Ognuno qui ha le sue sensibilità culturali e politiche, ma tutte sono convergenti affinché si possa dare finalmente, in questo scorcio di legislatura, un apporto che faccia anche presa su quella parte di Paese, che ormai è sfiduciato e che - ahimè - guarda, sì, al Parlamento ma in termini purtroppo negativi.

e dello sforzo collettivo che da parte di tutti i Gruppi è venuto nel lavoro in Commissione. Mi auguro che ciò sarà confermato anche dal voto dell'Assemblea, per giungere ad un testo più largamente condiviso su un provvedimento

e che costituiva l'elemento principale del suo disegno di legge, cioè la costituzione di un Comitato interparlamentare sui temi dello spazio, egli sa, perché ne abbiamo lungamente discusso anche nel corso del lavoro in Commissione, che noi abbiamo giudicato che quel tipo di istituzione (una Commissione interparlamentare)

politico-istituzionale delle politiche dello spazio e dell'aerospazio presso la Presidenza del Consiglio. Nel contempo, se posso dire, esso rischiava di confliggere anche con le competenze

alle Commissioni che lavorano su altri temi, come la difesa e così via. Insomma, ci sono già le istituzioni che possono fare il lavoro che il collega Bocchino

lo spazio - come abbiamo già detto in discussione generale - è un comparto strategico per il nostro Paese e per far sì che gli indirizzi politici vengano presi in conformità, non solamente delle politiche europee ma in

i compiti di indirizzo, coordinamento e direzione dell'intero settore con questo provvedimento sono attribuiti al Presidente del Consiglio, che, unitamente al Comitato interministeriale costituito, definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario, finendo per controllare l'Agenzia spaziale italiana, che perderebbe quindi molta dell'autonomia di cui gode oggi e che, a mio parere, è molto importante salvaguardare.

La *ratio* dell'emendamento è volta a garantire che il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, istituito presso presso la Presidenza del Consiglio, assicuri il coordinamento dei programmi e delle attività dell'ASI nonché delle società partecipate dall'ASI e, quindi, anche al CIRA. Come sapete, il Consorzio italiano di ricerche aerospaziali è una società consortile per azioni a maggioranza pubblica ed è sottoposto alla vigilanza del MIUR, al quale è stato affidato il compito, ai sensi della legge n. 184 del 1989, di dare attuazione al Programma nazionale di ricerca aerospaziale. Il CIRA però in questi ultimi anni ha subìto dei tagli che hanno compromesso notevolmente le attività di ricerca e per questo riteniamo sia fondamentale garantire una sua adeguata partecipazione per avere una sempre maggiore valorizzazione della ricerca aerospaziale. Il Governo dovrà adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire questa effettiva valorizzazione del CIRA, che si realizza, da una parte, attraverso il riconoscimento delle risorse necessarie e, dall'altra, con la rappresentatività. Per questo abbiamo presentato anche l'ordine del giorno G2.100, con il quale si intende impegnare il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire un'effettiva valorizzazione del CIRA, attraverso la destinazione di risorse umane e strumentali aggiuntive per la gestione delle attività caratteristiche, e a garantire un effettivo coinvolgimento del CIRA in quanto società partecipata dell'ASI nelle attività di programmazione coordinamento. È quindi necessario che il Governo si assuma la responsabilità di puntare sulla ricerca con delle iniziative concrete a supporto dello sviluppo del CIRA stesso e garantisca anche delle opportunità ai lavoratori del settore della ricerca che si trovano invece in una situazione di precariato. Maggiori risorse umane e maggiori risorse strumentali sono il minimo indispensabile per garantire la sopravvivenza del CIRA. Presidente, illustro gli emendamenti 2.107 e 2.109, che mirano ad introdurre, nell'ambito della decisione sui finanziamenti che farà questo Comitato governativo, anche la previsione di un programma obbligatorio di finanziamento della ricerca libera, il cui ammontare in percentuale sul totale degli investimenti è stabilito nella misura del 5 per cento, essenzialmente per tutelare la ricerca libera, appunto, che è basata sui satelliti e quindi sulle attività spaziali, in completa analogia - lo vorrei sottolineare doppiamente anche ai relatori - con quanto avviene con l'Agenzia spaziale europea, che fin dalla sua fondazione, per merito di Amaldi, uno dei suoi fondatori (tra l'altro italiano),

anche l'emendamento 2.116, che istituisce un consiglio di esperti per le politiche aerospaziali con funzioni consultive e propositive presso il Comitato, perché uno dei problemi che ha questo disegno di legge è proprio che l'aspetto consultivo e propositivo ed il coinvolgimento della comunità accademica ed industriale di questo Paese non sono previsti

promuove misure volte a sostenere la domanda e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali,

l'idea della *new space* con cui oggi ci confrontiamo non vede più al centro degli interessi della politica la conquista spaziale, ma riconosce nello spazio una nuova frontiera per la crescita lo sviluppo. Non è un caso che negli ultimi anni il numero dei Paesi e delle aziende che hanno investito in questo settore sia notevolmente aumentato, scatenando un'agguerrita competizione a livello internazionale. Dalla crisi del 2008, infatti, la media dei *budget* pubblici dei paesi OECD è scesa di pochissimo, passando da 52 a 50,8 miliardi di dollari nel 2013. Inoltre, sta emergendo anche il ruolo sempre più attivo, in questo settore, di nuove potenze come la Cina e l'India accanto agli Stati Uniti, alla Russia e al Giappone. La Commissione europea ha manifestato l'ambizioso obiettivo di collocare l'Europa in una posizione di *leadership* nel settore spaziale e aerospaziale anche se, al momento, gli investimenti europei nello spazio sono di poco inferiori ai 10 miliardi di euro. Nonostante ciò, il fatturato dell'industria spaziale europea è valutato tra i 47 e i 54 miliardi, occupando oltre 230.000 professionisti attivi anche nel comparto della produzione e dei servizi. Nel panorama europeo, l'Italia ha acquisito, negli ultimi anni, un ruolo di prim'ordine con un'industria spaziale che comprende circa 250 aziende e registra un fatturato complessivo di circa 1,6 miliardi.

il processo che ha permesso la nascita di una filiera industriale altamente specializzata e competitiva, tanto che oggi il nostro Paese è presente in tutta la catena produttiva legata allo spazio: satelliti, stazioni terra, lanciatori e analisi dei dati. Abbiamo, poi, alcune aziende di eccellenza che sono in grado di sfruttare i dati spaziali al servizio di applicazioni terrestri di pubblica utilità dal settore delle telecomunicazioni e della sicurezza a quello della salute e dei trasporti.

ricerca, nell'investimento e nel lavoro intorno a questa attività che può portare sicuramente qualcosa di buono, anche e soprattutto per il nostro PIL. La concorrenza dei Paesi emergenti come l'India

giunge all'esame dell'Assemblea dopo un *iter* che va avanti dal giugno 2014 e che ha visto non solo un ciclo di audizioni, ma anche la presentazione di diversi nuovi testi da parte Il provvedimento mira al riordino di un settore strategico per gli interessi del Paese con evidenti ricadute in termini di ricerca e di economia. Movimento democratico e progressista, vorrei ribadire alcune questioni che si ritengono molto importanti. Da un punto di vista strettamente giuridico, il testo non presenta particolari criticità. La questione che si pone, tuttavia, è di natura squisitamente politica, concernendo in particolar modo il tema dell'opportunità che i compiti di indirizzo, coordinamento e direzione dell'intero settore siano attribuiti al Presidente del Consiglio. Nello specifico egli, unitamente al costituito Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, approva il documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese; nonché finisce, sostanzialmente, per controllare l'Agenzia spaziale italiana, indirizzandola nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali. Si consideri che l'ASI oggi è un ente pubblico equiparato a qualsivoglia ente di ricerca e, per questo, è soggetto al Ministero dell'istruzione,

perderebbe molta dell'autonomia oggi a suo beneficio. Ci dispiace pertanto che non siano stati approvati gli emendamenti che a tale scopo avevamo presentato. Nonostante il grande lavoro svolto nella Commissione di merito, nel condivisibile obiettivo di costituire strumenti di *governance* nel settore dello spazio, si ritiene che si sarebbe dovuto maggiormente tutelare e garantire l'autonomia dell'Agenzia, anche sotto il profilo della sua discrezionale scelta

sulla strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini - la politica spaziale è sicuramente uno strumento importante per raggiungere obiettivi sociali, economici e strategici; sociali, per il benessere dei cittadini europei, che dipende molto dal progresso progresso tecnico-scientifico in tema di ambiente, di lotta ai cambiamenti climatici, di sicurezza e di sanità; economici, perché lo spazio genera nuove conoscenze ed è motore di innovazione, di crescita e, quindi, di posti di lavoro; strategici, perché una buona politica spaziale serve sicuramente a consolidare il ruolo dell'Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza politica ed economica. Voteremo, quindi, a favore, anche se ritenevamo importante definire meglio la funzione di raccordo del Comitato interministeriale tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali, per sostenere anche finanziariamente progetti capaci di avere positive ricadute sul territorio per quanto riguarda la crescita del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale. Votiamo, quindi, a favore, nella speranza che, in sede di attuazione, si tenga conto delle osservazioni fatte dal nostro Movimento.

Signor Presidente, arriva al traguardo un provvedimento che ha avuto un *iter* lungo non mesi, ma quattro anni, non mesi, ma quattro anni, e forse più. Se siamo qui oggi, lo dobbiamo al paziente e intelligente lavoro dei due relatori, la senatrice Pelino e il senatore Tomaselli, che ringrazio di cuore. Eppure, non eravamo sprovvisti di *governance*. È dal 1988 che ci siamo dotati di strumenti e di finanziamenti che hanno consentito all'Italia di essere

a quanto ha fatto il professore Broglio nell'ambito aerospaziale - era davvero nel gruppo di *élite* nel mondo. Oggi procediamo all'ammodernamento di questa *governance*, perché occorre sempre mantenere il passo con i tempi, in modo particolare in questi settori dove la ricerca e la tecnologia costituiscono la parte preponderante del lavoro richiesto per rimanere ai vertici mondiali. L'obiettivo dunque è chiaro e condividiamo il disegno di legge in esame, che intende costruire una politica spaziale e aerospaziale d'avanguardia, in un contesto economico e internazionale che - come si suol dire - è sempre più competitivo. Come dimostrano e insegnano le esperienze degli Stati Uniti, ma ora anche di altri Paesi che si stanno avvicinando o stanno maturando grandi interessi nell'aerospaziale, come la Cina, le ricadute delle politiche spaziali sulla vita non solo economica, ma anche civile e quindi dei cittadini, sono molto superiori a quello che può apparire a livello superficiale.

La relatrice Pelino ha detto che lo spazio va considerato come un sistema complesso per le conoscenze, i settori industriali, le applicazioni e gli utenti globalmente coinvolti e ha ragione:

la vita di tutti i cittadini. Pensiamo alle applicazioni nel campo dell'osservazione della terra, al miglioramento delle tecnologie e delle nanotecnologie e all'evoluzione dell'industria, che sono innegabili.

si annoverano circa 200 aziende, quasi 6.000 addetti, per una cifra che si avvicina ai 2 miliardi di euro di fatturato diretto.

difendere e sostenere la piccola e la microimpresa. Ma ricordiamo sempre che, se non c'è una filiera che parte da una grande impresa e da un grande disegno di strategia politica o di politica industriale, le piccole e le microimprese non possono svilupparsi, crescere e vivere. E, quindi, si genera una filiera che integra, mescola e collega tanti soggetti interessati al comparto spaziale. Con il disegno di legge in esame si vuole sancire la scelta multidisciplinare - riguarda i filoni dell'industria, dell'ambiente, dell'agricoltura, della difesa e dei trasporti

L'importanza del provvedimento si ricava poi anche dal fatto che alla fine la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche

la politica del settore. E il Comitato interministeriale avrà il precipuo compito di coordinare gli enti di ricerca e la pubblica amministrazione con il mondo dell'impresa. Ovviamente non c'è solo il tema delle ricadute economiche, che sono chiare, e della competitività del sistema nel suo complesso, ma c'è anche quello anche quello ricordato dai due ottimi relatori della sicurezza nazionale sia civile che militare; c'è il tema del raccordo con i programmi internazionali ed europei,

tutto ciò non mette in discussione l'azione dell'Agenzia spaziale italiana che, partecipando al Comitato interministeriale, diventerà il soggetto fondamentale di raccordo tra il sistema industriale e il mondo della ricerca. Ricordiamo anche che l'Agenzia italiana, per il prestigio acquisito e l'esperienza maturata, ha un ruolo di primo piano nei programmi dell'Agenzia spaziale europea.

anche allo sviluppo della Stazione spaziale internazionale. Per tali motivi il Gruppo Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa giudica opportuno e positivo il provvedimento e voterà a favore della nuova *governance* di politica spaziale e aerospaziale italiana. Signor Presidente, ho iniziato il mio intervento in discussione generale definendo questa giornata storica per il fatto che parliamo di politica spaziale in un'Aula parlamentare.

delle scelte fatte e rendendo in qualche modo trasparente il processo decisionale nel campo della politica spaziale. Per questo motivo noi non faremo mancare il nostro appoggio. Anzi, addirittura, riteniamo che la chiarificazione dei processi decisionali debba avvenire anche in altri campi come - ad esempio - in quello della ricerca. ricerca. Vi sono dei disegni di legge attualmente in discussione (uno a mia prima firma e uno a prima firma della vicepresidente Di Giorgi) che mirano, sostanzialmente, a istituire un comitato interministeriale per quanto riguarda la politica della ricerca. Anche la politica della ricerca, della quale la politica spaziale è - se vogliamo - un sottoinsieme, infatti, ha quei caratteri di multidisciplinarietà che fanno sì che i Ministeri coinvolti nelle decisioni siano

anche noi speriamo possa avvenire nel più breve tempo possibile, si possa continuare a discutere di politica spaziale in Parlamento, secondo alcune linee che riteniamo debbano essere affrontate

ancora formalmente un ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR pone una serie di problemi anche nel campo dei finanziamenti. In realtà, l'Agenzia spaziale italiana non è un ente pubblico di ricerca, ma un'agenzia, il vero e proprio braccio operativo del Governo nel campo della politica spaziale. Pertanto, abbiamo mancato l'occasione per strutturare meglio

il Comitato interministeriale dovrebbe nominare esso stesso

siffatta decisione un po' in antitesi rispetto a quello che succede in altre istituzioni scientifiche, come ad esempio negli enti pubblici di ricerca, dove questo comitato è, in parte o *in toto*, eletto dalla comunità scientifica, proprio perché deve essere la rappresentazione del contributo della comunità scientifica alla discussione delle politiche. Questa sorta di confusione fra i due ruoli permane anche nella definizione degli organi consultivi, con il risultato

per definire le linee lungo le quali il nostro Paese deve muoversi. Ritorno ancora una volta sul tema del coinvolgimento del Parlamento. La senatrice Pelino ha fatto cenno al fatto che

più importante di quello che ha attualmente. E questa è una discussione che abbiamo svolto tantissime volte in Aula, signor Presidente, quando si è parlato della riforma costituzionale, e che va fatta anche in siffatto campo. Ebbene, uno dei modi per far sì che il Parlamento torni ad avere il suo ruolo è anche quello di prevedere la possibilità, in materie interdisciplinari come queste - e quindi non ben rappresentabili e rappresentate dalle singole Commissioni parlamentari - di istituire un comitato che sorvegli e faccia un po' il cane da guardia nei confronti del Governo, nulla togliendo naturalmente alla facoltà e al potere del Governo di intervenire e decidere sulle grandi linee di indirizzo di politica spaziale. Sottolineo ancora una volta che si tratta di un'occasione persa, sulla quale dovremo ritornare. Ciononostante, per i motivi sopra detti, Sinistra Italiana non farà comunque mancare il suo appoggio a questo bell'intervento legislativo, atteso già da tanto tempo dagli operatori

Non nascondiamo, però, una piccola preoccupazione su alcune ambiguità e generalità di definizione, come quelle che si trovano nell'articolo 2, sullo sviluppo di programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare. Nonostante queste preoccupazioni, il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Colgo l'occasione per ringraziare la senatrice Pelino e il senatore Tomaselli per il lavoro svolto. svolto. È la dimostrazione, signor Presidente, che, quando il Parlamento lavora in maniera libera, i provvedimenti che escono da quest'Assemblea sono sicuramente migliori. Il Parlamento - secondo il mio modesto parere riprende quella centralità e quel potere che troppo spesso lascia al Governo di turno. Presidente, colleghi senatori, mi sia consentito innanzitutto ringraziare la senatrice Pelino per lo spirito e il lavoro che ha svolto nel portare avanti il disegno di legge in esame. L'industria aerospaziale riveste carattere strategico nelle economie avanzate, in quanto generatrice di ricchezza e di alte tecnologie, l'Italia, con i suoi due miliardi di euro, si posiziona al terzo posto in Europa dietro solo a Germania e Francia. Chi mi ha preceduto ha sottolineato come il ritorno economico delle attività di ricerca e applicazione tecnologica di questo settore siano di ben cinque volte superiori agli investimenti, con una concreta ricaduta sull'intero comparto industriale, perché dal settore aerospaziale derivano più brevetti e applicazioni che riguardano interi settori: dalle telecomunicazioni alla sicurezza, dalle infrastrutture alle costruzioni e persino alla farmacologia. Desidero sottolineare come il settore aerospaziale sia un'eccellenza italiana. Difatti, nonostante il nostro modello economico sia composto di una rete di medie e piccole industrie, si conferma all'avanguardia anche nei vari livelli che compongono la catena produttiva. E lo dimostrano i numerosi successi raccolti in questi anni nelle varie missioni spaziali a cui abbiamo contribuito mediante moduli abitativi, sistemi di comunicazione, satelliti scientifici e sistemi di propulsione. Si pensi alle numerose collaborazioni con la NASA, ormai consolidate negli anni, nonché alla nostra partecipazione con un ruolo primario all'ESA, Agenzia spaziale europea. Ed è proprio in ambito europeo che un'azienda italiana, la AVIO, ha fatto segnare l'ennesimo traguardo: la produzione del più grande motore monolitico in fibra di carbonio a propellente solido mai realizzato al mondo, che equipaggerà i nuovi lanciatori europei. Tuttavia, la grande dinamicità e l'efficienza delle nostre imprese non sono sufficienti a permettere al settore di dispiegare le potenzialità che realmente si possiedono. Serve infatti un'organizzazione unitaria e una politica industriale complessiva che impongano quelle risposte efficaci e quella visione strategica di cui il nostro Paese avrebbe un disperato bisogno, ma che gli ultimi Governi non sono stati in grado di garantire. Pertanto, il Gruppo Forza Italia non può che guardare con favore a un provvedimento che punta a dotare i settori spaziali e aerospaziali di un nuovo sistema di Governo che tenga sempre più presente la complessità delle sfide del comparto, la necessità di un approccio olistico garantito da un coordinamento strutturato e di ridare centralità al dibattito sul ruolo dell'industria spaziale in Italia; un compito fino a oggi egregiamente svolto dall'Agenzia spaziale italiana, che ha saputo guidare il settore rimanendo sempre all'avanguardia nel mondo, ma che ora sarà reso ancora più agevole grazie alla creazione di un comitato di coordinamento, posto sotto la direzione e la responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei Ministri, che possa efficacemente affiancare l'ASI. Per sottolineare la reale inversione di tendenza e la centralità che si intende dare al tema delle politiche aerospaziali è sufficiente scorrere l'elenco dei Ministri previsti da questo provvedimento nel Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale: dieci Ministri a cui si aggiungono il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e il Presidente dell'Agenzia spaziale italiana. Alla luce di quanto appena esposto e nella speranza che il percorso intrapreso per il settore aerospaziale con questo disegno di legge, mediante la definizione di strategie, politiche industriali, sinergie e linee di sviluppo, possa rappresentare la strada maestra da seguire per lo sviluppo dell'intero Paese con una politica industriale degna di questo nome,

dei principali interventi legislativi per garantirne uno sviluppo sempre maggiore. Il settore aerospaziale ha ad oggi profonde e significative ricadute anche in termini strettamente economici e di crescita del nostro Paese: non è più soltanto uno straordinario settore di ricerca e di sperimentazione, ma rappresenta ormai una irrinunciabile ed effettiva opportunità di sviluppo economico e sociale. Molti risultano essere i campi in cui si palesano gli effetti prodotti dalla ricerca aerospaziale attraverso l'applicazione concreta del frutto della ricerca nel tessuto sociale del Paese. La molteplicità delle applicazioni è vastissima e diversificata, estendendosi dall'astrofisica e dalla cosmologia al monitoraggio dei cambiamenti climatici, alla sicurezza (inclusa la gestione dei disastri naturali), alla difesa, al trasporto, all'agricoltura, all'ambiente marittimo, alle previsioni meteorologiche, alla società dell'informazione, alla salute, all'energia e *smart cities*, al mercato delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare, per citare alcune delle possibili applicazioni. È cresciuta, dunque, l'importanza del valore socio-economico del settore aerospaziale, come ampiamente rappresentato anche nel corso delle audizioni e nelle relazioni introduttive ai disegni di legge in discussione, che hanno evidenziato l'esponenziale e significativa crescita del numero di Paesi con capacità spaziali nel mondo. A ciò si aggiunga lo sviluppo che ha avuto il settore in Italia (come precedentemente richiamato anche dal relatore) con la nascita, in varie Regioni, da Nord a Sud, di veri e propri distretti economico-produttivi, che vedono la numerosa presenza di aziende di piccole e medie dimensioni, che sono essenziali per alimentare il ciclo produttivo delle grandi imprese che operano in questo campo. A livello italiano, solo per fornire qualche dato numerico, si calcola che l'economia legata allo spazio rappresenti un giro di affari di 1,5 miliardi di euro nell'anno 2014. Ma si può fare molto di più molto di più ed è con questa convinzione che il Governo ha istituito innanzitutto una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui partecipano l'Agenzia spaziale italiana

all'istituzione di un Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Come avete detto, il Comitato avrà il compito di indirizzare e supportare l'Agenzia spaziale nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con i diversi soggetti internazionali definendo quindi il prospetto delle risorse finanziarie da impiegare. Avrà il compito di promuovere i processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, nonché lo sviluppo ed il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese e, cosa sicuramente non meno importante, i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità (ambiente, trasporto, telecomunicazioni). Si calcola, a tal proposito, che un euro investito nel settore dello spazio diventi poco più nel caso in cui l'investimento verta sul settore scientifico, cosa comunque necessaria per aumentare la conoscenza e sperimentare nuove tecnologie, ma addirittura a fronte di un euro si può arrivare a sei euro in ambiti particolarmente remunerativi come quello delle telecomunicazioni. Questo per dire dell'importanza, anche in termini economici, di questo settore. materia peraltro è innegabile, posti le conoscenze, i settori industriali, le applicazioni, gli operatori e gli utenti globalmente coinvolti, nonché il numero molto elevato di cooperazioni e *partnership* internazionali. settore, oltre ad essere espressione d'eccellenza tecnologica in chiave strategica, soprattutto con funzioni di deterrenza e di accrescimento del prestigio, rappresenta oggi un importante traino per il rafforzamento della competitività industriale del Paese. Fattori abilitanti di tali opportunità sono le capacità industriali, risultato di scelte di una politica industriale che oggi più che mai è importante in uno scenario sempre più globale, ma anche sempre più affollato di concorrenti, mira ad assicurare la competitività di un sistema industriale che sia in grado, da un lato, di servire la domanda istituzionale, e, dall'altro, d'imporsi e affermarsi con profitto nel mercato commerciale internazionale. Con favore, quindi, durante i lavori è stata accolta la necessità di riformare il mandato dell'ASI, ponendo maggiore attenzione allo sviluppo industriale del comparto spaziale nazionale, con particolare riferimento anche ai bisogni della grande, della piccola e della media impresa. È importante quindi che le soluzioni di *governance* *in fieri* possano sviluppare il tessuto connettivo intorno all'Agenzia, affinché, da un lato, questa continui la propria missione nell'ambito della ricerca e del rafforzamento della competitività industriale

Per tutti i motivi che ho qui sommariamente riportato e con l'auspicio che il settore dello spazio e dell'aerospazio possa essere oggetto di costante e crescente attenzione da parte del legislatore e del Governo, il Gruppo del Partito Democratico voterà convintamente a favore del disegno di legge che ci accingiamo a votare.

una prospettiva eccezionale sono lavoratori che lavorano attraverso un *software* che vendono oggi anche all'estero. Ebbene, cosa vogliono fare?

non ha assolutamente senso, vista anche la tipologia di lavoro che svolgono. Voglio allora chiedere al Ministro di intervenire affinché questo non accada e i lavoratori

con questo intervento di fine seduta continuo, oggi, al Senato, una staffetta con cui, assieme a tante senatrici e tanti senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è o è stata legata da relazione amorosa. Lo faremo fino a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne. Il 14 maggio, a Castel Volturno, in provincia di Caserta, è morta Binta Sani, di a seguito delle ferite da accoltellamento riportate, tre giorni prima, nel tentativo di difendere un'amica dall'aggressione del suo ex compagno. Il 18 maggio a Trebaseleghe, in provincia di Padova, una donna di quarantasei anni, Natasha Bettiolo, è stata uccisa a coltellate dall'uomo con cui aveva una relazione. Dopo averla uccisa, l'uomo ha tentato il suicidio. Salgono così a 57 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno 2016. Ricordo, inoltre, che dopo due anni di indagini, ieri, 23 maggio, è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale, il marito di Angela Della Torre, quarantanove anni, di Castellabbate, in provincia di Salerno, morta a seguito di una spinta ricevuta durante una violenta lite. Il femminicidio è solo la punta dell'*iceberg* della violenza maschile nei confronti delle donne. In Italia sono oltre 8,3 milioni le donne vittime di violenza psicologica e 4,5 milioni quelle quelle che hanno subito atti sessuali degradanti e umilianti, rapporti non desiderati e subiti come violenza, abusi o molestie fisiche sessuali. C'è ancora un enorme lavoro da fare per estirpare dalla nostra società il cancro della violenza sulle donne. Ci deve essere un grande impegno educativo e culturale soprattutto verso le giovani generazioni, a partire dalle scuole. Va fatto conoscere il fenomeno, in tutti i suoi tragici risvolti, e va promossa una campagna contro ogni forma di violenza e per promuovere e radicare la cultura del rispetto. Riproponiamo con convinzione il nostro appello. Un appello al Governo tutto e alla Sottosegretaria con delega alle pari opportunità: la cabina di regia monitori l'applicazione, i pregi e i limiti della legge n. 119 del 2013, e soprattutto dia piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Un appello ai *media*: si smetta di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. Un appello agli uomini e alle donne di questo Paese: sono state più di centoventi le donne uccise nel 2016; non possiamo più accettare questa mattanza. *(Applausi